saranno poste ai voti le dimissioni presentate dai senatori Giaretta e Danieli. Comunico all'Aula che, poiché la seduta si concluderà alle ore 13, alle ore 12,45 si voteranno le due dimissioni. Comunico altresì che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata a conclusione della seduta antimeridiana, per stabilire, in particolare, la data di discussione delle comunicazioni che il Governo renderà al Senato sulla politica estera.

Signor Presidente, onorevoli senatori e senatrici, innanzitutto desidero ringraziarvi per il lavoro svolto in queste settimane

In merito alla discussione che si è svolta, mi preme semplicemente specificare un elemento. Mi pare corretto sottolinearlo, anche

e dotandosi di strumenti che possano dare una risposta concreta al bisogno delle famiglie. Affinché ciò possa avvenire, però, è necessario - questo è il secondo punto che volevo sottolineare

per consentire sia un monitoraggio del fabbisogno di abitazioni necessarie sul territorio italiano, sia la progettazione di interventi per migliorare l'offerta di alloggi con affitto a basso costo. Sottolineo questo elemento, perché è del tutto evidente che la situazione in cui ci troviamo registra, sulla questione della casa, una vera e propria emergenza. Si tratta di un problema che ha difficoltà ad assumere dignità politica,

tanto che il numero di sfratti per morosità è in continua crescita. Credo che il punto che abbiamo di fronte questa mattina è certo quello del blocco degli sfratti per le categorie svantaggiate - cosa giusta

calmieratore del mercato, né di intervenire positivamente per dare una risposta alla necessità di case e al diritto all' abitare delle fasce sociali più deboli. più deboli. Altri Paesi europei, con Governi di vario colore, hanno dimostrato un'attenzione al tema della casa di tutt'altra natura. Il Governo francese ha dato vita ad un piano che prevede la costruzione di 150.000 nuovi alloggi all'anno per sei anni,

anche al fine di decidere le forme e i modi attraverso cui stanziare risorse da parte dello Stato, per favorire il processo di ripresa di una politica pubblica sulla casa. casa. Vi ringrazio per il lavoro compiuto e credo che l'approvazione di questo disegno di legge sarà salutata positivamente da molte migliaia di famiglie per di famiglie per l'ossigeno che offre nella gestione di problemi molto pesanti come quello degli sfratti per fine locazione per le categorie svantaggiate.

per l'individuazione del fabbisogno e la conseguente individuazione delle risorse finanziarie, che permetta al Governo, insieme alle Regioni che ne hanno la titolarità, di predisporre una politica pubblica per

per i beneficiari del credito di imposta di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 106 del 2005, esprime parere non ostativo, ad eccezione che sull'articolo 9, comma 2, sul quale il parere è contrario, attesi gli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento sul 2008, derivanti dalla conservazione in conto residui delle somme indicate a copertura del provvedimento e atteso che, pur prendendo favorevolmente atto della volontà del Ministro di dar corso positivo alla richiesta di conservazione in bilancio dei residui, il relativo procedimento amministrativo per l'iscrizione dei medesimi nel bilancio 2007 risulta avviato ma non ancora completato. Osserva poi quanto segue: - la quantificazione degli oneri indicata nella relazione tecnica relativa ai benefìci fiscali previsti dall'articolo 2, fa riferimento a dati risalenti all'anno 2003 e non risulta aggiornata ai dati più recenti ancorché disponibili; - il meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'articolo 9, comma 2, del disegno di legge, non appare conforme alla legge di contabilità di Stato, sia per quanto attiene all'impiego di risorse di conto capitale sia per la copertura di oneri di parte corrente, non apparendo idoneo il transito in tesoreria per la modifica della natura degli oneri. Esprime parere non ostativo su tutti gli emendamenti, ad eccezione che sugli emendamenti 1.4, 1.10, 2.1, 4.0.1 e 1.100, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

e ripropone il testo del disegno di legge, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori del Gruppo Forza Italia in materia, evidenziando così come il Gruppo Forza Italia ha alla sua attenzione l'argomento, ma non può condividere l'estensione

alla dizione originaria per cui sono state concesse nel tempo molte proroghe, ma mai nessuna di estensione temporale o di fattispecie, riducendo l'intervento nei Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti, piuttosto che estenderlo a quasi tutto il territorio nazionale. Allo stesso modo, con la demagogica parvenza del discorso sociale, che poi si riduce di molto nelle cifre dallo stesso Governo indicate, quando abbiamo giustamente approvato la pregiudiziale di costituzionalità sul decreto-legge del Governo, che introduceva elementi con pareri addirittura contrari ai sensi dell'articolo 81 da parte della stessa Commissione bilancio, si è scatenata una gara al «dalli all'untore» su questo argomento, dicendo che volevamo bloccare gli interessi di milioni di famiglie. La stessa relazione del Governo riconduce in termini quasi

La necessità di ricondurre la norma ad una effettiva esigenza sociale ma di non introdurre elementi surrettizi è espressa anche dall'emendamento 1.42: 1.42: laddove, così come poco fa ha detto il Ministro, estendiamo la possibilità di usufruire della proroga *ope legis* alle famiglie che hanno figli fiscalmente a carico, introduciamo una platea

che presiedono alle esigenze del disagio abitativo. Ancora una volta, utilizzando un tema socialmente importante, si vuole invece intervenire a danno di una categoria,

La soppressione del comma 3, che proponiamo con l'emendamento 1.44, torna su una delle motivazioni, signor Presidente, che abbiamo

Comunque, la soppressione del comma 3 in questione si impone per le stesse motivazioni per cui fu approvata la pregiudiziale del 25 ottobre 2006. introduce una differenza di trattamento tra soggetti beneficiari a seconda delle qualità, non dell'inquilino, quindi delle condizioni soggettive di disagio abitativo, ma del concedente, attraverso una differenziazione tra concedenti, se siano piccoli proprietari o grandi enti. Si introduce allora un meccanismo di differenziazione del privilegio concesso della proroga ai titolari degli stessi requisiti. Vi è di più.

le caratteristiche dei soggetti beneficiari di tale disposizione. Lo stesso Ministro, poco fa, ha accennato a una volontà interpretativa.

che le norme siano formulate male e poi abbiano bisogno di interpretazioni. Siamo in una sede parlamentare e abbiamo il dovere di correggere le norme formulate male per dare chiarezza ai cittadini che debbono utilizzarle e comprendere chi abbia diritto Ora, la dizione: «anche indirettamente, svolgono l'attività di gestione dei relativi patrimoni immobiliari, il termini di sospensione di cui al comma 1...» è inequivocabile: si riferisce al termine di sospensione, non alla qualità dei soggetti beneficiari. Occorre pertanto specificare, aggiungendo alla fine del comma 3 le seguenti parole: «fermi restando i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al medesimo comma 1»; diversamente, la norma si potrebbe rendere applicabile a tutti coloro che occupano immobili posseduti da queste società. Quindi, alla palese violazione costituzionale della differenza di trattamento, si aggiungerebbe addirittura una contraddizione in termini nel dare accesso a una sospensione dei provvedimenti di sfratto di 18 mesi a chiunque, senza tener conto della situazione di disagio abitativo.

delle percentuali e constatiamo che possono rientrarci anche quelle categorie.

quei soldi possono essere amplificati con l'edilizia agevolata che ha un moltiplicatore 15 rispetto ai fondi posizionati nella norma. Ancora, possiamo vendere i patrimoni degli ex IACP sui quali lo Stato spende milioni, miliardi di euro per la manutenzione, laddove si pagano affitti che vanno fino a 5-10 euro mensili.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta discutiamo il provvedimento di interventi per la riduzione del disagio abitativo facendo particolare attenzione

non soltanto degli enti o delle casse di previdenza ma anche di coloro i quali sono proprietari di 100 appartamenti di trovare un'altra casa con un minore assillo. Questo provvedimento deve, una volta per sempre, dare la possibilità che per il futuro non si debba ancora rinviare gli sfratti e dare sempre maggiore preoccupazione a quelli che si trovano in particolari situazioni di disagio sociale. Mentre la Francia provvede con un provvedimento a costruire ogni anno 150.000 appartamenti per sei anni, noi ci riempiamo soltanto di parole. Mi auguro che tutte le promesse che sono state fatte oggi dal Governo non siano vuote parole ma servano a risolvere il problema delle abitazioni in Italia.

che qui non si tratta solo, sotto alcuni profili, di valutare la giustizia, l'equità e, diciamo, il *favor* per le categorie più disagiate del provvedimento - che potrebbe in astratto trovarci trovarci consenzienti anche in misura più larga -; si tratta di valutare anche la compatibilità di questa normativa con la nostra Carta costituzionale e con la giurisprudenza della Corte costituzionale. dopo anni e anni di tirate d'orecchie al Parlamento, ha finalmente dichiarato illegittime le norme in materia, proprio sulla base di alcuni principi che hanno fatto scuola per la legislazione futura, cioè principi abbastanza ben delineati che devono servire come guida per interventi di questo tipo. Ora, noi abbiamo contestato che ci sia questa aderenza della norma all'articolo 1, in molti punti, a questi princìpi, in particolare,

in quest'Aula, che venisse fornito l'elenco dei Comuni, il combinato disposto di questa normativa che unisce i capoluoghi di provincia e i Comuni limitrofi con almeno 10.000 abitanti con i Comuni ad alta densità abitativa, per vedere quale è la mappatura, che indubbiamente è ampliata, e di moltissimo, rispetto agli ultimi interventi che hanno caratterizzato questa materia. alla questione della durata della proroga, al comma 3 di cui è stato detto, che riguarda i cosiddetti grandi proprietari, cioè gli enti pubblici (che poi hanno dei conti economici da equilibrare), si prevede una proroga di diciotto mesi che è esorbitante rispetto alle necessità funzionali alla soluzione di questi problemi che devono essere considerati, risolvibili in termini più brevi, come è previsto, tra l'altro, nella norma di carattere generale di cui al comma 1 dell'articolo 1. Mi fa piacere per altro, signor Presidente, lo devo dire, che il Ministro - credo con interpretazione autentica - abbia risolto quel dubbio sull'ultimo periodo del comma 1, in base al quale poteva sembrare che l'estensione della proroga della sospensione degli sfratti riguardasse le famiglie con un certo numero di figli a carico prescindendo dagli altri requisiti; che di questa dichiarazione sia preso atto e che costituisca, insieme a quella resa anche dal relatore e nel dibattito dell'Aula, un mezzo per evitare che si apra a dismisura la portata di questa normativa e che quindi possa impattare con i princìpi costituzionali espressi dalla Corte che ho brevemente citato.

noi saremmo per chiedere a tutti i presentatori degli emendamenti di ritirarli, in virtù della necessità di una approvazione rapida e definitiva di questo provvedimento legislativo, ricordando anche - ma loro lo sapranno - che questo disegno di legge è già stato approvato alla Camera dei deputati con larga maggioranza. Nel merito, abbiamo già risposto nella replica e lo ha ribadito anche il signor Ministro poc'anzi, per cui, ove i presentatori degli emendamenti dovessero insistere per il loro mantenimento, il parere su tutti è un parere contrario.

la stessa necessità di arrivare con urgenza all'approvazione del disegno di legge fa sì che la discussione nel merito degli emendamenti, per quanto mi riguarda, passi in qualche modo in secondo piano, perché c'è un problema di urgenza. Su alcuni, altrimenti, esprimerei un consenso, su altri un dissenso. Per quanto riguarda il Governo, il problema fondamentale è arrivare ad una approvazione rapida, vista la situazione critica presente nelle città.

che il disegno di legge in esame è lontano dal nostro pensiero federalista. È inutile che da Roma si vogliono regolare le tensioni abitative su tutto il Paese.

il Governo avrebbe dovuto dirci quanti sono stati gli sfratti eseguiti dall'ultima proroga sino ad oggi per motivare l'urgenza. La cifra sarebbe stata contenuta in pochissime decine

estremamente ampia platea di soggetti beneficiari. Stiamo intervenendo per legge in rapporti contrattuali tra le parti e quindi abbiamo la necessità di ridurre

riconduce la materia nei termini di tutte le precedenti proroghe che hanno sicuramente interessato i veri centri dove si possono verificare fenomeni di disagio abitativo ed in particolare le grandi città.

dal nostro Gruppo, il quale intende che questo provvedimento eccezionale sia limitato solamente alle grandi città, dove effettivamente esiste un disagio abitativo, fermi restando i requisiti soggettivi dei beneficiari.

Signor Presidente, già nel corso dell'illustrazione ho evidenziato i motivi dell'opportunità di eliminare il comma 3 dal testo introduce una forte differenziazione tra gli stessi soggetti beneficiari, in virtù della qualità di di colui che dà in affitto l'appartamento. A parità di diritti si introduce una differenziazione tra coloro che sono soggetti alle norme del disagio abitativo.

perché nella parte finale del comma si fa riferimento al termine di sospensione previsto dal comma 1 e non già ai requisiti soggettivi che danno diritto alla proroga. Per come è genera sicuramente confusione perché tutti coloro che attualmente sono inquilini di questa tipologia di proprietà - dunque le grandi società, le proprietà derivanti dagli ex enti previdenziali e quant'altro - possono avere diritto a questa maxi proroga.

tutti coloro che attualmente sono inquilini delle grandi società, in buona parte derivantida ex istituti previdenziali - lo sappiamo perché ne abbiamo denunciati a iosa di episodi di affittopoli negli anni passati - si possono «acquattare» dietro questa norma ottenendo una proroga delle condizioni di assoluto vantaggio delle quali, indebitamente e senza avere

*(FI)*. Signor Presidente, sono veramente molto sorpreso delle motivazioni assolutamente pretestuose per cui si nega qualsiasi modifica a questo testo. Sappiamo benissimo, per esperienza ormai consolidata, che quando vi è la cosiddetta volontà politica (qui pare che vi sia, perché anche parte dell'opposizione inspiegabilmente segue una deriva demagogica con l'obiettivo di approvare oggi questo provvedimento), nel giro di 24 ore nel giro di 24 ore - l'esperienza ci insegna - si restituisce il testo alla Camera dei deputati e lo si approva. Lo abbiamo fatto per tantissime norme, sia con questo Governo che con i precedenti. Non

l'individua - dell'opportunità politica. Quindi, il nostro Gruppo si asterrà sull'articolo 1, a fronte dell'ostinata presa di posizione del Governo e del relatore, i quali impediscono al Parlamento di valutare le proposte emendative al disegno di legge con la sola scusa

sta votando sistematicamente contro le modifiche di questo testo, contro modifiche assolutamente logiche e assolutamente limitative dell'invasività di una norma sui rapporti contrattuali dei cittadini. Questo è un Governo che sbandiera liberalizzazioni, ma ma difficilmente troveremo nella storia del Parlamento, in questa materia, una proroga che entra così pesantemente, «a piedi uniti», sulla libertà contrattuale Attenzione quando ci si ammanta di determinate qualifiche: bisogna essere sempre coerenti quando si assumono atteggiamenti e indirizzi politici tesi a liberalizzare i rapporti tra i cittadini nella nostra società.

si verificherà sull'intero disegno di legge. Noi stessi abbiamo presentato un disegno di legge in materia, ma sul vero disagio abitativo e non utilizzando il disagio abitativo come cavallo di Troia per entrare in numerosissimi rapporti, con un'estensione territoriale e sociale che va

intervengo soltanto per dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale. Al collega senatore D'Alì voglio dire che ci sono dei passaggi nei disegni di legge o nei decreti‑legge che si possono condividere o meno. Il nostro Gruppo ha compiuto una valutazione evidentemente

che in quest'Aula si sia dimostrato, in altre occasioni, che il Gruppo di Alleanza Nazionale sia in qualche modo connivente con questo Governo: non lo credo assolutamente. Questo è un provvedimento di carattere sociale che noi condividiamo: lo voteremo e lo difenderemo fino in fondo

la mia presa di posizione di sopprimere l'articolo 4, sulla concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica, Ci sono grandi storie sull'edilizia residenziale pubblica: e il nostro Paese sarebbe bene ne venisse a capo una volta per tutte e non sicuramente con questo articolo.

rimandare il più vicino possibile alle persone le decisioni sull'abitazione:

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

per capire quale possa essere la motivazione per cui il Parlamento, in particolare la Camera, e il Governo nella proposizione del testo si siano orientati ad entrare *ope legis* nei rapporti contrattuali tra cittadini, dove il disagio abitativo non c'entra nulla. Quindi, per prima cosa questo è un articolo che non ha niente a che vedere con il titolo della legge. In secondo luogo, questo articolo, se i colleghi non lo avessero letto attentamente, prevede una modifica sostanziale di rapporti contrattuali liberamente stabiliti tra le parti. Potrei comprendere che, se si volesse innovare la normativa che regola i fitti degli esercizi commerciali, si potrebbe anche immaginare una norma che ha effetto per il futuro, non certo effetto retroattivo. Ci siamo battuti per anni perché i rapporti tra i cittadini cittadini e tra Stato e cittadini (vedi lo statuto del contribuente) non avessero effetti retroattivi e le norme non intervenissero a piè pari sulla libertà contrattuale dei cittadini.

mi sembra veramente paradossale. Se vi sono dei casi specifici che meritano di essere presi in considerazione da singole istituzioni, da Comuni o dallo stesso Ministero per i beni culturali, si intervenga *ad adiuvandum* nell'azione dei conduttori, ma non certo a penalizzare la proprietà dei locatori; e non si intervenga generalizzando su tutto il territorio nazionale le motivazioni, che possono pur essere legittime, di un singolo caso. Questa è una di quelle leggi leggi che anche la sinistra, allora opposizione, amava definire fotografia e che poi si applicano all'intero territorio nazionale. Allora, con maggiore onestà intellettuale si sarebbe potuti entrare nello specifico di alcuni eventuali casi autorizzando i Ministeri o le istituzioni competenti a intervenire a sostegno di un'attività, non a penalizzazione di altra attività con una norma che coinvolge l'intero Ma l'abbiamo letto bene questo articolo 7? Questo significa autorizzare il Parlamento nel caso specifico a intervenire su un numero «n» di casi esistenti esistenti sul territorio nazionale, introducendo nuovamente in queste Aule parlamentari un principio che abbiamo lottato per condannare, quello dell'ingerenza dello Stato nei rapporti tra i cittadini. Infatti, se oggi tocca alle attività teatrali,

È chiaro, tutti ci facciamo cogliere dalle tentazioni dirigiste in questo Parlamento. Il giorno in cui avrò il piacere di incontrare un autentico liberale forse stapperò una bottiglia di *champagne*.

potrebbe essere estesa a tante altre categorie. Ma ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo dal punto di vista concettuale? Non voglio entrare nel merito della singola fattispecie, ma dal punto di vista generale stiamo modificando per legge rapporti liberamente stabiliti tra cittadini contraenti. Se questo è il principio che vogliamo affermare, noi siamo fermamente contrari.

di indicarci quanti sono stati i casi in cui l'urgenza è venuta meno dal 25 ottobre fin ad ora per cui oggi la si invoca disperatamente. Ci sono altre motivazioni che sottendono a tale necessità e noi non possiamo condividerle.

perché condivide il testo dell'articolo 7 e gli obiettivi cui tale articolo si propone di pervenire. di pervenire. Mi esprimo con grande serenità e con la pacatezza che credo mi si debba riconoscere ha sempre contraddistinto i miei interventi in Aula e nelle Commissioni: non accettiamo l'accusa del senatore D'Alì di voler condividere un provvedimento dirigista e vogliamo rassicurarlo del fatto che, almeno per quanto ci riguarda, non siamo disponibili a un provvedimento che, come lui indica, intervenga «a gamba tesa» indiscriminatamente nei rapporti fra cittadini e nei rapporti contrattuali.

anche ottusa e miope, senza badare alle ragioni contrastanti che il legislatore ha sempre l'obbligo di bilanciare. Si è spesso detto della nostra presunta saggezza nell'esercizio delle nostre funzioni: questa è un'occasione.

con l'emendamento 7.100. Ci sono ragioni precise che il senatore D'Alì o non è stato in grado di intendere o non ha voluto intendere e che io desidero illustrare all'Aula perché ne sia rassicurata. Abbiamo pensato ai cinema e verificato che il saldo dei posti offerti agli italiani dall'industria cinematografica dopo la chiusura delle sale storiche ma dopo l'apertura di numerose nuove multisale è positivo:

La prima osservazione che mi viene in mente ma che certamente non poteva essere ospitata nel provvedimento legislativo in esame, di cui rivendico la necessità di approvazione senza rinvio alla Camera, è quella di riservare a una competenza regionale, provinciale o comunale la definizione del

Il numero dei proprietari di botteghe storiche è assolutamente incontrollabile nell'intero territorio nazionale e si riferisce anche a singoli proprietari di singoli immobili. Viceversa, nel caso del teatro, si sono verificate e si verificano queste condizioni: una straordinaria perdita di posti offerti, per usufruire dell'attività teatrale, ai cittadini, attraverso le progressive chiusure in tutte le città; una perdita pluriculturale, perché chiudere i teatri non vuol dire semplicemente privarsi dell'attività artistica degli attori, ma anche di coloro che scrivono i testi

di persone - lo dico tra molte virgolette - raggiunte dal provvedimento in termini per loro non favorevoli. Ecco la capacità che il legislatore deve avere di saper mediare tra i i diritti e le opportunità e le possibilità che devono essere offerte ai cittadini; ecco la saggezza che il legislatore deve avere nel saper anche fare un passo indietro rispetto alle direzioni principali che ha per sé stabilito. Per Alleanza Nazionale restano quelle liberistiche; in questa occasione è viceversa condivisa un'operazione come quella che il disegno di legge propone, quindi il voto su questo emendamento sarà contrario, come pure sui successivi.

perché l'articolo 7, un articolo estemporaneo rispetto al contesto del provvedimento, il quale ultimo, tra l'altro mantiene un titolo insufficiente rispetto alla portata che esso ha assunto con l'approvazione alla Camera dello stesso articolo 7 (delle cui vicende siamo naturalmente a conoscenza), pone problemi molto delicati di merito ma soprattutto di legittimità costituzionale, Presidente, come abbiamo rilevato anche in Commissione affari costituzionali e come accennato nel parere reso

mantenendo soltanto alcuni comparti senza però allargarli più di tanto, a tutela sociale, a tutela magari delle attività commerciali, a tutela delle attività alberghiere. Ricordo che per gli alberghi da tempo immemore vi è una normativa vincolistica, che man mano si è liberalizzata, però si è mantenuto per gli alberghi il termine di durata contrattuale dei nove anni più Quindi, il testo dell'articolo 7 va in contraddizione con la linea politica consolidata nella legislazione italiana. In secondo luogo, questo testo - ciò che è più grave

In base a quale ragione costituzionale, in base a quale norma degli articoli 41 e 42 della Costituzione, riteniamo che il tipo di esercizio o di attività degli immobili destinati a teatri sia di tale rilevanza sociale, di tale impatto sociale, di tale utilità pubblica da determinare un'entrata nei contratti in corso e penalizzare i proprietari che magari, fidando nella durata del contratto (che non è poco, sei più stanno organizzando un diverso modo di disporre dell'immobile di cui sono legittimamente proprietari? Questo è il punto più forte. Sono convinto che, ancorché questo testo sia stato dettato e approvato sembra - per un caso singolo, e non nascondendo la rilevanza che può avere a livello nazionale, genererà sicuramente contenziosi a non finire, perché questa norma è palesemente incostituzionale. poi, queste ragioni sociali devono essere portate avanti e realizzate dalla mano pubblica, non a carico di questo o quel proprietario che per ventura si trovi ad

vorrei rassicurare gli amici che hanno parlato a favore di questo articolo sul fatto che grande è la nostra sensibilità per i problemi del teatro. Vogliamo appoggiare il teatro? Vogliamo sostenere con più forza l'attività teatrale in Italia? Sì, certamente, ma a spese della fiscalità generale, non riversando l'onere della solidarietà su alcuni cittadini scelti a caso, e non si capisce bene perché lo debbano sostenere loro e non altri per il semplice fatto che casualmente sono proprietari degli immobili sui quali insiste quel determinato contratto. Aggiungerò ma non vorrei ripetere quello che ha detto così bene il senatore Pastore - che interveniamo in contratti in corso, violiamo l'autonomia delle parti. lo Stato è titolare di un diritto primario diretto d'intervento sulle botteghe artistiche, o è campo che in termini costituzionali è assegnato, alla luce della riforma costituzionale realizzata, piuttosto alle Regioni, se non addirittura ai Comuni? Siamo in grande imbarazzo perché, al di là dell'articolo 7, tutto questo provvedimento mantiene un conflitto di due valori costituzionali: uno è il diritto all'abitazione, l'altro è il diritto alla libera disponibilità della proprietà ed anche il diritto all'equità, perché non solo nel caso dei teatri, ma in generale, un dovere di solidarietà che noi sentiamo concretizzato, poiché la casa è un dritto, viene scaricato su una categoria di cittadini i quali non hanno, a parte il fatto casuale di essere proprietari di quegli immobili, nessun elemento di vantaggio che porti a dire che loro sono i più ricchi, i più forti e quindi è giusto che portino quel peso. In molti casi, sono più deboli di tanti altri soggetti che hanno fatto investimenti diversi e proprio per questo non vengono penalizzati da parte dello Stato. Mi auguravo che, seguendo una linea legislativa che da tempo sta cercando di portare equità in questo campo, si responsabilizzassero le Regioni per far fronte alla tensione abitativa, magari si fosse un po' più generosi nel dar loro risorse, ma si provvedesse, come si fa in tutti Paesi europei, ad affrontare il tema senza mettere in contrasto fra di loro i diritti di alcuni con i diritti di altri. Ancora una volta, invece, daremo soddisfazione, giustamente, ai diritti di alcuni, ma penalizzeremo, ingiustamente, i diritti di altri. dopo l'intervento del senatore Buttiglione sarò brevissimo, perché ha detto esattamente quello che io per altro sosterrò - insisto - nella dichiarazione di voto con particolari che il

contro cittadini inermi, grazie a questo Parlamento che fa provvedimenti populisti. Ma lo dimostrerò con i fatti nella mia dichiarazione di voto.

vuole esprimere la propria perplessità in ordine a questo punto del provvedimento, che ci sembra non congruo con le finalità e risponda sicuramente a una storia e a una preoccupazione legittima.

Presidente, voglio ricordare ai colleghi che sull'articolo 9 vi è il parere contrario della 5ª Commissione, anche se semplice (cioè non ai sensi dell'articolo 81 Il parere contrario, però, è importante, perché va a intercettare una prassi che è sempre stata negata, nella nostra storia parlamentare, sulle leggi di bilancio,

I motivi per cui cadde il decreto-legge sul disagio abitativo, presentato dal Governo in quest'Aula il 25 ottobre 2006, furono proprio legati alla copertura finanziaria dello stesso provvedimento o all'espressione di un parere negativo da parte della 5ª Commissione.

onorevoli colleghi, a distanza di qualche mese ci troviamo nuovamente in quest'Aula a discutere l'annosa questione della proroga degli sfratti. Come Come tutti sanno, la questione può ormai dirsi più che datata perché abbiamo assistito, nell'ultimo ventennio, con cadenza quasi annuale, a continue reiterazioni di questa tipologia di intervento.

con cadenza quasi annuale, a continue reiterazioni di questa tipologia di intervento. A quanto pare, a nulla valgono le continue ammonizioni pervenute sia dalla Corte costituzionale che, più recentemente, dalla Corte di cassazione, le quali ci ricordano che il legislatore, pur dovendo farsi carico delle esigenze di coloro che si trovano in particolari condizioni di disagio, non può limitarsi a trasferire all'infinito l'onere relativo, in via esclusiva, a carico del locatore, che è un cittadino come gli altri, che spesso rappresenta la fascia debole nel rapporto tra locatore e inquilino e potrebbe trovarsi egli stesso in identiche situazioni di disagio. La sospensione degli sfratti, in sostanza, può trovare giustificazione soltanto se incide sul diritto alla riconsegna dell'immobile per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato. A nostro giudizio, poco vale che in questo disegno di legge si sia introdotta una specifica norma che apparentemente tutela il proprietario che si trovi in condizioni di disagio simili al proprio inquilino. è che queste continue reiterazioni hanno finito per trasformare quelli che dovevano essere provvedimenti transitori in una disciplina quasi ordinaria a scapito e a danno di un'intera categoria sociale, quella dei proprietari di immobili. A loro danno e a loro scapito c'è la prassi: ormai nei tribunali civili la decisione è sempre in favore dell'inquilino. Noi non siamo insensibili alla pesante situazione in cui si trovano a dover vivere molti cittadini, ma non possiamo non ricordare in quest'Aula e in modo particolare qualora non li avesse presenti, alcuni princìpi cardine del nostro ordinamento, come quello della proprietà privata e i diritti ad essa connessi, che, al pari di tutti gli altri qui oggi invocati, risulta tutelata dalla nostra stessa Costituzione. Se spogliamo il concetto di proprietà da quello di godimento del bene, priviamo lo stesso del suo contenuto essenziale. Poche parole ancora, signor Presidente. Oggi abbiamo una nuova categoria di disagiati che proprio questo dirigismo parlamentare ha creato;

Come nella precedente discussione che ha investito il decreto presentato dal Governo, noi ribadiamo con fermezza che la soluzione ad un così grave disagio sociale, come quello legato all'abitazione, non può in alcun modo essere riversata sui privati cittadini, resi colpevoli di aver potuto, anche a costo di gravi sacrifici, acquistare un'abitazione. Queste continue reiterazioni hanno portato all'esasperazione e generato angoscia in buona parte della categoria dei proprietari, ma i problemi non si limitano a ciò. Tale esasperazione, infatti, induce, a causa di una tortuosa reazione a catena, alla produzione di molteplici effetti negativi. Non si possono biasimare tutti quei proprietari che ben si guardano dal mettere sul mercato degli affitti il proprio immobile nel timore di non poterne mai più usufruire. È una legittima difesa! Ciò a sua volta genera un'inevitabile contrazione del mercato degli affitti, soprattutto nelle grandi città, e quindi la lievitazione dei costi. Noi tutti sappiamo, poi, come si evolve e degenera ci troviamo di fronte ad ulteriori fenomeni che investono la nostra società e che riguardano in modo particolare i giovani, i quali non possono più permettersi di andare via dalla casa dei genitori, le giovani coppie, che faticano a trovare un'abitazione idonea alle proprie necessità, o ancora le famiglie con reddito medio, che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Qualora poi questo disegno di legge dovesse superare anche l'esame del Senato, non potremmo fare a meno di paventare ulteriori rischi. Il Governo ha, infatti, legato alla soglia dei 27.000 euro di reddito la possibilità di usufruire di tale blocco. Noi ci domandiamo a buon diritto se non si è tenuto conto del forte incentivo, costituito dalla soglia di 27.000 euro, all'evasione fiscale, fenomeno già di vaste proporzioni nel nostro Paese. Intere categorie sarebbero così portate a rimanere all'interno di questa soglia in modo da poter, tra l'altro, beneficiare di tale blocco a scapito di chi, invece, ha probabilmente sempre pagato le proprie tasse. Non si possono dimenticare, infatti, i dati elaborati dall'erario

di reddito e, ancora più stranamente o - oserei dire - assurdamente, emergerebbe che i gioiellieri e i titolari di bar dichiarano al fisco meno dei 21.500 euro dei maestri elementari ad inizio carriera, o risulterebbe che i proprietari di saloni per la vendita di autovetture di Piemonte, Lazio e Campania denunciano un reddito inferiore ai 16.000 euro, cioè un reddito inferiore a quello dei loro concittadini che da quindici anni varcano il portone di Mirafiori, Cassino e Pomigliano d'Arco come metalmeccanici. Sotto i metalmeccanici sarebbe anche la media dichiarata dai tassisti. Quindi, avete compreso che fra quegli inquilini si nascondono fasce di privilegio che al contrario dobbiamo colpire, mentre dobbiamo agire come Stato, come Regioni e come Comuni, facendoci carico noi e non altri cittadini che si trovano nelle medesime condizioni dei disagi delle fasce più deboli.

Il Governo ha previsto la possibilità di evitare il blocco per quella categoria di proprietari che si trovi nella stessa situazione di bisogno degli inquilini, ma non prevede

Forse ci scordiamo la media dei tempi dei giudizi nei nostri tribunali. Questi proprietari, già esasperati dai continui blocchi, dai tempi biblici della nostra giustizia, vedranno ulteriormente rinviata la possibilità di riavere il proprio immobile poiché nulla si stabilisce sui tempi massimi che i giudici dovranno dare per produrre l'idonea documentazione e conseguentemente per il rilascio dell'immobile. Si potrebbe arrivare, così, al paradosso che molti proprietari troveranno non conveniente usufruire dell'esenzione, con l'unica paura che, allo scadere di quest'ulteriore periodo, il blocco verrà ancora una volta - ed è probabile, se non cambia la coscienza di questo Parlamento - reiterato. A questo punto ci chiediamo: avrà mai termine quest'emergenza? Arriveremo al punto in cui si trasferirà automaticamente la proprietà di questi immobili agli affittuari bisognosi? La strada potrebbe praticamente sembrare questa. Ma non è sicuramente l'unico paradosso di questo disegno di legge. Se il Governo ritiene che la soglia dei 27.000 euro sia idonea a stabilire che un nucleo familiare si trovi in uno stato di necessità tale da giustificare il sacrificio imposto a un'altra famiglia, per quale motivo pretende contemporaneamente, dalla stessa famiglia bisognosa, il versamento delle tasse? Non sarebbe più logico equiparare tale soglia a quella di esenzione dalla tassazione o innalzare quest'ultima e, quindi, caricare sullo Stato tali necessità e non a un altro privato? Insomma, la normativa sul blocco degli sfratti è da sempre palesemente iniqua - mi avvio alla conclusione, Presidente - soprattutto se si tiene presente che altrettanta solerzia e incisività non è dedicata a tutelare quelle centinaia di migliaia di famiglie che da anni lottano per riavere il proprio immobile, frustrate dai tempi della giustizia. Questi cittadini non hanno altrettanti diritti? Perché non si agisce con polso fermo sulla grave situazione degli immobili di proprietà degli istituti di case popolari, abusivamente occupati da generazioni da falsi bisognosi? Perché non si prevedono misure realmente efficaci per favorire l'acquisto della propria abitazione? Perché non si cerca di individuare misure strutturali alternative che consentano al Governo di poter svolgere la propria funzione sociale senza liberarsi del fardello a scapito dei cittadini stessi? Perché un Governo che ha scontentato tutti con le sue liberalizzazioni indiscriminate, invece di reiterare il blocco, non liberalizza definitivamente anche il mercato degli affitti? Basta tribunali, avvocati, lungaggini assurde, ma solo incentivi sotto forma di sgravi fiscali ed esenzioni dall'ICI per quei proprietari che immettono sul mercato degli affitti immobili, magari a lungo termine o con possibilità di rinnovo per giovani coppie, *single* o per famiglie disagiate, senza il timore di rimanere private per un tempo indeterminato dei propri beni. dei propri beni. Temporeggiare ulteriormente non risolverà questa che non è più un'emergenza, ma un cancro che si diffonde nel nostro Paese da molti anni. È finito il tempo dei provvedimenti passivi. È ora che ci si faccia carico della situazione mettendo in campo azioni concrete e risolutive.

nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Verdi‑Comunisti italiani e Consumatori uniti al disegno di legge, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni.

Innanzitutto, vorrei ricordare che il provvedimento, al contrario di quelli che lo hanno preceduto nella scorsa legislatura, non affronta solo e unicamente l'emergenza;

decreti che non facevano altro che prorogare il termine di esecuzione degli sfratti: punto e basta. Questa era la realtà che abbiamo trovato. Ciò accadeva

i dati del fabbisogno degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e soprattutto una ricognizione della situazione nel nostro Paese. nostro Paese. Vorrei ricordare che questo elemento è fondamentale anche per la gestione della contingenza degli sfratti. Si torna finalmente, con elementi di novità apprezzabili,

in capo ai Comuni, ma ovviamente coordinate dai Prefetti. Altro elemento fondamentale è l'istituzione del tavolo di concertazione finalizzato a definire un programma nazionale di edilizia residenziale pubblica. Credo sarà l'occasione non solo di contemperare gli interessi, ma di cominciare a comprendere come si è evoluto il fabbisogno abitativo nel nostro Paese, quali sono gli elementi di crisi e anche come deve evolversi

non ci sono soltanto i classici piani di edilizia residenziale pubblica, c'è la possibilità di incrementare - e il nostro Gruppo è estremamente favorevole - anche le politiche di recupero.

piano dà in mano ai Comuni, ai Ministeri e alle Regioni la possibilità concreta di comprendere come contrastare il fenomeno, che in questi anni è stato impressionante, del *boom* immobiliare, che

affitti. Dovrebbe essere nella sensibilità di quest'Aula comprendere che è arrivato anche il momento di cominciare a rimetter mano alla legge n. 431 del 1998, perché essa non è più rispondente agli elementi di novità subentrati in questi anni nel mercato immobiliare. Contemporaneamente, lo sottolineava giustamente il Ministro, abbiamo avuto una drastica riduzione della proprietà pubblica nel campo degli alloggi, anche a causa del fenomeno della cartolarizzazione.

complessivo familiare. Contemporaneamente, queste stesse norme e condizioni si applicano anche al conduttore, qualora dovesse venire a trovarsi in queste condizioni.

in enti previdenziali, casse professionali e società assicurative, che rappresentano nei Comuni a grande disagio abitativo il nocciolo duro

È il primo provvedimento per ricominciare a costruire in modo serio, dopo anni di nulla, una politica di Governo per l'abitazione. Ho

Signor Presidente, membri del Governo, sono pienamente consapevole che nel Paese Italia ci siano situazioni di disagio abitativo, ma di certo non si può pensare che tale disagio si possa risolvere con una legge centralista come quella al nostro esame. Il mio pensiero federalista convinto e continuo

L'idea di normare tutto con dei numeri non può essere condivisa, laddove invece la nostra idea è di avere cittadini con pari diritti.

a disposizione di portatori di *handicap,* si vede invece ridicolizzato quando un giorno, per necessità personale o di nuclei familiari, non può poi eseguire uno sfratto, magari anche concordato, perché l'inquilino non solo è portatore di *handicap*, ma non ha una sufficiente entrata che gli permette di trovarsi di trovarsi un'abitazione magari sullo stesso territorio ma in un'altra proprietà. Questa situazione ricade

Il nostro movimento - che mi sento fortemente onorato di rappresentare - ha un forte senso di solidarietà, così diffuso nella nostra terra. È bello quel proverbio milanese che dice «Chi gira ul cú a Milan a gira ul cú al Pa». Sant'Ambrogio nel Trecento aveva fatto capire che vi era questo grande spirito di solidarietà nel popolo padano, che vediamo ancora adesso diffuso su tutto il territorio, su tutto il Paese Italia, fortemente sensibile, e che ci ha resi così nobili nella storia del nostro Paese. Dunque, giusto perché abbiamo così forte il senso di solidarietà nella nostra terra e nel nostro popolo, l'idea di un voto contrario su questo provvedimento

stancherò mai di invitare il Governo ad un processo federalista nella gestione del nostro Paese. Abbiamo Abbiamo parlato di prima Repubblica, e di seconda Repubblica, ma il senso importante della trasformazione di uno Stato centralista e centralizzato come questo ne può venir fuori, nella sua situazione di rinnovamento del mondo della politica, solo percorrendo la strada federalista. Mi auguro che quanto prima il Governo ponga attenzione a questo senso della politica. Dunque, annuncio il voto del Gruppo che mi onoro di rappresentare, che sarà un voto di astensione.

appare evidente la necessità di un provvedimento volto a ridurre il disagio abitativo soprattutto nelle grandi Città in considerazione della situazione che si è venuta a determinare alla scadenza della precedente proroga; data in cui hanno riacquisito la loro efficacia i provvedimenti di sfratto. Un Governo nato in nome dell'equità e delle liberalizzazioni stava varando un provvedimento inaccettabile. Il disegno di legge in esame oggi, pur con vari miglioramenti, mostra molte lacune e pone alcune problematiche, i cui effetti potrebbero determinare un aggravio di oneri per lo Stato; innanzitutto, la sussistenza dei presupposti costituzionali del disegno di legge in questione viene smentita da grandi dubbi di incostituzionalità di alcune disposizioni, come si desume dalle più recenti sentenze della Corte costituzionale, secondo le quali le politiche sociali non possono essere realizzate a danno di alcune componenti della collettività. Proprio per rispettare tale principio, nella scorsa legislatura il Governo aveva istituito un fondo destinato a sostenere le politiche di contrasto al disagio abitativo. Contestiamo l'articolo 1, comma 1, che estende in misura irragionevole a tutti i capoluoghi di Provincia e ai Comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti la sospensione delle procedure esecutive di rilascio. Abbiamo parlato a lungo del problema del disagio abitativo delle grandi Città; con questo provvedimento abbiamo esteso indiscriminatamente la platea di coloro che ne subiscono gli effetti. Il Governo deve fornire,

Ci lascia dubbiosi anche il successivo comma 3, che proroga, con un termine maggiore, le sospensioni riguardanti gli immobili di casse professionali e previdenziali, compagnie di assicurazione, istituti bancari e società immobiliari, determinando una procedura esecutiva di rilascio in base alla condizione soggettiva non già del conduttore, bensì del locatore. Tale disposizione determina un'immotivata disparità di trattamento, prevedendo una proroga più lunga per i conduttori di immobili di cui siano proprietari alcuni particolari enti. Non abbiamo avuto i necessari chiarimenti sulla copertura finanziaria della norma di cui all'articolo 2, che autorizza i Comuni a prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili a favore dei locatori danneggiati dalla sospensione delle procedure di sfratto. L'articolo 4, che prevede la definizione di un piano pluriennale nazionale straordinario di edilizia residenziale pubblica, rappresenta certamente un disegno strategico per affrontare la questione abitativa, ma tale piano non può essere costretto nell'ambito di un provvedimento che consideriamo di urgenza, per questo ci lascia perplessi. Non dimentichiamo che le competenze sono già in capo alle Regioni, che spesso sono poco sensibili, salvo lamentarsene poi con lo Stato. Crediamo da sempre nella necessità di varare norme che prevedano e agevolino la possibilità di acquisto della casa da parte di tutti, principalmente da parte di persone in situazioni particolari, da parte delle giovani coppie che, come sapete bene, è inutile ripeterlo anche oggi, hanno problemi enormi e spessissimo decidono di non formare una famiglia, non perché non vogliono ma perché i problemi reali sostanziali giornalieri sono troppi e tanti e questo è sicuramente il principale. Rischiamo, caro Presidente, di cadere come sempre nelle chiacchiere e in politica le chiacchiere rischiano sempre di rimanere tali. È evidente l'incongruità in generale delle norme che prevedono la predisposizione di programmi pluriennali, come dicevo, di edilizia sovvenzionata e agevolata da parte dei Comuni, senza però provvedere alle necessarie risorse. Crediamo,

Ci siamo impegnati con nostre proposte e continueremo. Crediamo, signor Presidente, che il nostro dovere sia quello di fare buone leggi, che non solo risolvano i problemi ma li prevengano; leggi che guardano avanti. Oggi, ancora una volta, siamo guidati dall'emergenza, un'emergenza purtroppo viziata dall'ideologia. Per questo motivo, consapevoli dell'emergenza, ma anche delle ideologie che viziano questo lavoro, oggi il Gruppo dell'UDC si asterrà.

anche nella replica di stamattina, la questione. Abbiamo la consapevolezza, e di questo il Governo ha dato atto, che si tratta di un intervento urgente, di emergenza,

pubblica, fa sì che il crollo dell'attività edificatoria dell'edilizia sociale, cui ha fatto riferimento stamattina il ministro Ferrero, sia drammatico

che perdono il diritto all'abitare. Mi rendo conto che ci può essere un danno economico nelle aspettative di un proprietario di alloggi,

operazioni di patrimonio cartolarizzato. Ma voi conoscete i casi di coloro i quali perdono l'identità di cittadini perché hanno perso il diritto alla casa, perché hanno perso l'alloggio? Conoscete i casi di impiegati pubblici che dormono nelle macchine parcheggiate agli angoli delle strade

con 90 famiglie senza casa, senza tetto, con bambini, e ha dichiarato che in quel palazzo intende realizzare il ministero dell'abitare, non perché pensi

ma perché intende sottolineare la necessità e l'urgenza di definire e realizzare un piano di edilizia residenziale pubblica che nelle condizioni di oggi,

gli elementi importanti di questa legge non sono tanto il giusto provvedimento di sospensione degli sfratti esecutivi, rispetto ai quali - devo dire la verità - ho trovato e trovo quotidianamente maggiore sensibilità da parte dei prefetti e delle autorità locali e da parte delle forze dell'ordine che vengono chiamate ad assistere l'ufficiale giudiziario di quanta non ne abbia avvertita qui dentro, in quest'Aula, da parte di alcuni interventi. Una sensibilità sociale che in quegli operatori c'è, e invece, nel distacco e nella subordinazione al diritto di proprietà rispetto al diritto all'abitare, non ho sentito in quest'Aula.

l'articolo 4 perché si definiscono - mi pare in termini opportuni - un programma e un progetto, che è quello della concertazione di un programma con le Regioni e con gli enti locali, l'individuazione di obiettivi e di indirizzi anche insieme alle Regioni, facendo salvo salvo qualsiasi elemento di specificità e di federalismo - se di questo si vuole parlare - e con proposte normative in materia fiscale adeguate. Un rapporto che non può che essere di cooperazione efficiente tra Stato e Regioni, ma dove un piano ha come primo compito, come primo dovere dovere da imporre a sé stesso quello di essere realizzato, di non rimanere lettera morta, di non restare un programma presentato bene, ma che non ha poi possibilità di realizzazione. Da questo punto di vista, sappiamo che ci sono le condizioni per destinare risorse pubbliche sia per costruire programmi integrati tra il pubblico e il privato capaci di garantire l'edilizia sovvenzionata per le fasce più deboli e la politica di accoglienza, sia per fare quelle politiche abitative legate al canone al canone convenzionato e alla realizzazione di alloggi da destinare all'affitto permanente per garantire proprio quella mobilità dei cittadini di cui tanto si parla.

che è in discussione per la beatificazione, ha affrontato il problema nella sua città e all'Isolotto di Firenze prevedendo e attuando la requisizione quando c'era il problema di dare la casa ai suoi cittadini fiorentini. Sarebbe bene che molti sindaci seguissero quell'esempio di fronte al dramma nelle loro città.

ero giustificato. Signor Presidente,colleghi senatori, la casa è un diritto affermato dalla Carta universale dei diritti dell'uomo, un diritto per i cittadini al quale corrisponde il dovere istituzionale per chi governa di adoperarsi per il suo rispetto, in special modo a tutela di particolari categorie di soggetti svantaggiati, che vivono nel quotidiano il peso gravosissimo del disagio abitativo. Proprio in relazione a tale dovere, il Governo ha responsabilmente emanato un disegno di legge che ripropone i contenuti del decreto-legge n. 261 del 2006, non convertito in legge a seguito dell'approvazione, da parte del Senato, di una questione pregiudiziale. Si prevede, proprio al fine di contenere il suddetto disagio abitativo, la sospensione per un periodo di otto mesi dell'esecuzione dei provvedimenti fondati sulla finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ma non quelli per morosità. Regola ispiratrice del testo è il sostegno per categorie sociali particolarmente svantaggiate, individuate in funzione di criteri oggettivi quali il reddito, un familiare fiscalmente a carico ultrasessantacinquenne, figli portatori di*handicap*, familiari con malattie terminali. Dunque, con l'approvazione del disegno di legge in questione, che ha superato il passaggio alla Camera con il costruttivo contributo dell'opposizione, a dimostrazione che su questioni importanti, di drammatica tensione sociale, è ben possibile trovare un proficuo accordo, si impedirà che in città come Roma, Milano e Napoli, in città capoluogo di Provincia e in città confinanti con oltre 1 milione di abitanti, nonché nei Comuni con alta tensione abitativa, operino brutali procedure di sfratto. Degne di menzione, poi, sono le disposizioni contenute all'articolo 2, che prevede il riconoscimento di benefici fiscali per i proprietari degli immobili locati, subito in conseguenza del mancato rilascio dell'immobile. Con questa previsione si è ottemperato a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 155 del 2004, nella quale la Corte aveva rilevato che l'onere del diritto all'abitazione gravasse ingiustamente solo sui locatori. Concludendo, annuncio a nome dei Popolari-Udeur il voto favorevole al provvedimento in oggetto, che affronta in termini costruttivi il problema del disagio abitativo, con la certezza che il Governo, nei prossimi mesi, adotterà soluzioni di sistema tese a raggiungere l'obiettivo di normalizzare il mercato delle locazioni, cercando di

la vicenda che oggi affrontiamo con questo disegno di legge, ed è una storia assai risalente, tuttavia, nel tempo. Negli interventi che vi sono stati nel corso della discussione generale e per l'illustrazione e poi il voto degli emendamenti,

Essenzialmente, vi sono state due posizioni della Corte che si sono succedute nel tempo: la prima è stata quella di accompagnamento, di sostegno, di favoreggiamento, in qualche maniera, di una politica che è andata avanti dalla metà degli anni '70 in maniera eclatante, prima in maniera derivante, di scivolamento, di blocco assoluto delle esecuzioni. Questo ha portato, per esempio, a plurime condanne del nostro Paese sul piano e europeo e ha portato anche ad ulteriori e non secondarie conseguenze. sulla base di questa difesa ad oltranza di quel sistema da parte della Corte costituzionale si è in qualche maniera seduta

usciva definitivamente dal controllo di chi ne era proprietario, per essere anche arbitrariamente utilizzata da chi ne aveva la locazione attraverso un contratto di locazione. Questo ha determinato una straordinaria conflittualità che tutti noi abbiamo conosciuto e che ricordiamo perfettamente. Alla straordinaria conflittualità sono derivati due tipi di reazioni:

nostra economia. Peggiore è la reazione, viceversa, di coloro i quali avevano in affitto le case che, consapevoli del fatto di godere di un privilegio che non sarebbe potuto durare a lungo, hanno inseguito il mercato immobiliare con una tendenza all'acquisto che, nel nostro Paese, è la più elevata di tutta Europa e non commensurabile rispetto - per esempio - agli Stati Uniti. Il che è per un certo verso un bene, perché assicura una abitazione in proprietà ad un grandissimo numero di concittadini ma, per altro verso, determina due conseguenze da valutare che affido alla vostra sensibilità. La è di tipo squisitamente ambientalistico: vi è stata una occupazione indiscriminata del territorio, peraltro spesso affidata ad esecuzioni immobiliari di scarso profilo e quindi tendenti ad un utilizzo

dei pesi che il nostro Paese è stato ed è ancora chiamato a dover sopportare. C'è stata poi una seconda fase della Corte costituzionale la quale, con una virata di 180 gradi, ha più volte richiamato il legislatore ad intervenire in maniera organica nel sistema ed ha determinato la legge di riforma delle locazioni, che ha reso quello che oggi è un mercato sostanzialmente libero un mercato sostanzialmente libero in cui, tuttavia, si introduce la necessità di azioni anche legislative di accompagnamento verso un definitivo regime. Oggi ci troviamo di fronte ad una legge che è indispensabile in questa logica, perché realizza quel principio di mediazione, che prima richiamavo intervenendo su un emendamento, con riferimento non solo ai soggetti più deboli, signor Presidente, ma anche alle situazioni più drammatiche.

ritiene che questo avvenga per sottolineare una profonda differenza che esiste tra il testo contenuto nel decreto-legge e quello contenuto nel disegno di legge oggi al nostro esame. Ho parlato del concetto di mediazione. Perché vi sia mediazione, occorre conciliare opposte necessità ed opposti diritti. Ho parlato dei soggetti più deboli e delle situazioni più drammatiche, che sono l'una categoria. Se andiamo a vedere l'altra categoria, ritorno a sottolineare la differenza esistente tra il decreto-legge che decadde perché non sostenuto nei presupposti di costituzionalità dalla maggioranza e dal Governo e questo disegno di legge. La differenza sta nel fatto che nel disegno di legge mancano, tra coloro i quali sono chiamati a sopportare l'onere della mediazione - mi esprimerò in questa maniera - i «soggetti» - leggo testualmente - «fisici o giuridici titolari di oltre 100 unità immobiliari ad uso abitativo, anche se diffuse in tutto il territorio nazionale». So bene che, anche nel

Si dice, infatti, che soggetto passivo di quella mediazione non sono coloro i quali, possedendo un immobile in forma fisica o in forma giuridica, costituiscono un'impresa non vi è discriminazione di mercato tra l'impresa che commercia frutta e quella che commercia immobili, il che rappresenta, signor Presidente, un passo fortemente innovativo in questo settore - ma

ma semplicemente di garanzia per la tutela dei patrimoni, nell'interesse di tutti i

ma - l'ho spiegato prima e lo ribadisco ora - un'emergenza culturale: e noi anche di cultura desideriamo continuare a vivere in questo Paese.

a danno di altri cittadini; credo che anche questo, se - com'è stato fatto, almeno per quanto mi riguarda, in maniera ponderata - non costituisce un gravame per molti, sia mediazione e possa essere accettato. Il Gruppo di Alleanza Nazionale, signor Presidente, voterà a favore di questo disegno di legge. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia si asterrà su questo provvedimento, che a nostro giudizio avrebbe potuto essere largamente migliorato se il Governo e la maggioranza fossero usciti dalla logica dell'urgenza.

lesivo di più norme fondamentali del nostro modo di operare. Il senatore Barbato poco fa - forse inavvertitamente - ha dichiarato di essere a favore del provvedimento

Su questo punto torno a chiedere con insistenza alla Presidenza di far sapere quando la questione verrà trattata nella Giunta per il Regolamento, così come il presidente Marini, con cortese nota inviatami, mi ha assicurato, quando ho sollevato il problema. Per il resto, confermiamo tutte le perplessità su un provvedimento che di buono ha il titolo - ed è per questo che anche noi ci eravamo impegnati nel presentare un nostro disegno di legge omonimo - ma che di assai preoccupante ha molte parti del suo contenuto, per cui ci asterremo

Signor Presidente, colleghi, un Parlamento, quando si trova a riproporre, con imbarazzante ritmicità, una proroga di deroga a proprie leggi, sta dichiarando la difficoltà se non l'incapacità - di individuare la soluzione del problema. Sul tema - è stato già ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto - è persino intervenuta più volte la Corte costituzionale per per dichiarare la improponibilità di questa reiterazione di deroghe. La legge n. 431 del 1998 aveva profondamente innovato il mercato dell'affitto liberalizzandolo e introducendo numerose tipologie contrattuali. L'introduzione del Fondo sociale per il sostegno dell'affitto, utilizzato da 400.000 nuclei familiari, si era rivelato strumento prezioso per alleviare il disagio abitativo. Il passaggio del patrimonio di edilizia popolare alle Regioni, accompagnato dalle modifiche del Titolo V della Costituzione, aveva l'obiettivo di responsabilizzare le istituzioni più vicine ai cittadini. C'era, in sostanza, una politica per la casa. Dobbiamo riconoscere, invece, che nei cinque anni trascorsi non vi è stata né la prosecuzione di queste politiche né una organica politica sulla casa, fosse anche di segno contrario. Si è impoverito progressivamente il patrimonio immobiliare pubblico con le operazioni di cartolarizzazione, sottraendo una quota importante di immobili ad affitto concordato. Si è nettamente ridotto l'impegno nella realizzazione di alloggi di edilizia pubblica, fino ai risibili 1.900 appartamenti del 2004. Si è ripetutamente decurtato il Fondo sociale per il sostegno dell'affitto, rendendo più complicato per gli enti locali aiutare i nuclei familiari più bisognosi, nel mentre si proclamava ad alta voce di appoggiare politiche a sostegno della famiglia. Le dinamiche economiche del periodo dell'ultimo quinquennio hanno portato ad un rilevante incremento del valore degli immobili e, conseguentemente, degli affitti. Ci siamo quindi trovati di fronte ad una condizione come quella odierna, in cui abbiamo 600.000 famiglie nelle graduatorie per gli alloggi di edilizia pubblica. Ad aggravare il disagio c'è l'importante flusso di stranieri, prevalentemente extracomunitari, che ormai assommano a 2 milioni e mezzo di cittadini, di cui circa un milione versa in condizioni di particolare disagio o di pauroso affollamento abitativo e di selvaggia speculazione, come del resto è stato dimostrato e denunciato da recenti tragedie verificatesi proprio qui a Roma. È quindi indispensabile approvare questo provvedimento per bloccare gli sfratti e alleviare, se non risolvere, il problema del disagio almeno per le famiglie più bisognose e che si trovano nelle particolari condizioni previste dal provvedimento stesso. Va ricordato, però, che ci si è preoccupati anche di ridurre il disagio per i proprietari di immobili, che oggi sono sullo stesso piano dell'affittuario e che ricevono agevolazioni fiscali e l'incremento del 20 per cento dell'affitto. A questo proposito, va sollecitato il provvedimento di cui si è spesso parlato negli ultimi tempi, che, nell'ambito della necessaria armonizzazione delle aliquote sulle rendite finanziarie, porti all'equiparazione della rendita da locazione a quella finanziaria. Va inoltre sottolineato - mi si perdonerà questo riferimento un po' polemico che pur apprezzando il positivo approccio odierno di Alleanza Nazionale e in parte di tutta la Casa delle Libertà a questo provvedimento, non possiamo dimenticare che in nome di un'effimera vittoria di tattica parlamentare si è riusciti a perdere quattro mesi nei quali alcuni sfratti - sia pure pochi, grazie anche all'azione del Ministro dell'interno - sono stati eseguiti. Ne sono derivati gravi disagi a nuclei familiari già tanto in difficoltà. Non possiamo però illuderci che questo provvedimento possa essere l'ultimo. Abbiamo sottolineato tutti la positiva presenza dell'avvio di una fase di concertazione e programmazione che prevede il coinvolgimento, in uno con il Governo, di Regioni, enti locali e organizzazioni rappresentative di inquilini e proprietari. Ma sappiamo altrettanto bene che la soluzione non è disponibile in tempi brevi. brevi. Ricordo che mediamente trascorrono, tra programmi e realizzazioni, in questo campo, circa sette anni. C'è quindi bisogno di politiche innovative. Tutti conveniamo sul fatto che l'edilizia pubblica, così come l'abbiamo conosciuta, è da ritenersi superata. È necessario il coinvolgimento dei privati ed il reperimento di adeguate risorse finanziarie. È anche chiaro che vanno individuati strumenti fiscali che liberino e mettano a disposizione del mercato quella parte non trascurabile di patrimonio immobiliare oggi inutilizzato, come pure andranno riattivati i programmi di recupero e di riqualificazione del patrimonio immobiliare delle città (penso alla legge obiettivo per le città). C'è, quindi, ancora tanto da fare. Questo è un primo, importante e positivo passo e, per tale motivo, il Gruppo dell'Ulivo voterà a favore del provvedimento

la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sulle dimissioni presentate dal senatore Giaretta. I senatori favorevoli ad accogliere le dimissioni premeranno il tasto verde al centro della postazione di voto; i senatori contrari premeranno il tasto rosso a destra; i senatori che intendono astenersi premeranno il tasto bianco a sinistra. Poiché si tratta di uno scrutinio segreto, qualunque sia la scelta di voto effettuata, la luce che si accenderà sarà di colore neutro.

Danieli. Pregherei i colleghi di stare seduti al proprio posto, evitando di porre giornali sopra le schede eventualmente utilizzate per il voto.

Per favore, vuole stare seduto, senatore Garraffa! Ci sono due senatori qui che svolgono le funzioni di segretari, rispetto ai quali lei non ha il diritto di sostituirsi! *(Vivi applausi